Signor Presidente, il gruppo francese Michelin è, come noto, *leader* mondiale nella produzione di pneumatici per tutti i tipi di veicolo, è presente con 68 siti di produzione nei cinque continenti e con un fatturato consolidato al 2008 di circa 16.400 miliardi di euro. In Italia, il gruppo è presente sin dal 1907 e possiede quattro stabilimenti di produzione situati ad Alessandria, Cuneo, Stura (in provincia di Torino) e Fossano (in provincia di Cuneo). In particolare, lo stabilimento di Stura produce pneumatici per autovetture di media e piccola cilindrata e tessuti gommati tessili e metallici. A tal riguardo, occorre evidenziare che nel mercato degli pneumatici piccoli e medi, le esportazioni in Europa da parte di costruttori asiatici sono aumentate notevolmente. In questo segmento di mercato il prezzo del prodotto diventa sempre più fattore determinante nella scelta dei clienti. Il contenimento dei costi di produzione risulta, dunque, vitale nella concorrenza tra i produttori. Il sito di Stura, in particolare, pur avendo realizzato nel corso del 2008 notevoli recuperi di produttività e di costo, deve rapportarsi con una realtà concorrenziale estremamente agguerrita costituita da produttori dei Paesi *low cost*. La grave situazione di crisi economica che sta travolgendo i mercati mondiali ha, ulteriormente, evidenziato le criticità del mercato dei pneumatici sopra descritte. In tale contesto, la Michelin ha presentato alle organizzazioni sindacali un piano di riorganizzazione delle sue attività in Italia, finalizzato a consolidare la propria presenza nel territorio nazionale. Tale piano prevedeva in sintesi: l'investimento di 200 milioni di euro nel quinquennio 2009-2013; la concentrazione nel sito di Cuneo della produzione di pneumatici vettura entro fine 2009; il trasferimento del magazzino di Vercelli a Torino Stura, entro i primi mesi del 2010, e l'ampliamento e il rafforzamento del ruolo di coordinamento della sede centrale di Torino; la creazione nel sito di Stura, entro la fine del 2010, di un importante centro logistico denominato SMA (Super Magazzino Amont) per lo stoccaggio e lo smistamento dei pneumatici destinati al mercato del rimpiazzo. I lavoratori interessati dal piano industriale sono circa 600 a Stura, 40 ad Alessandria e 40 Vercelli, dove la società possiede uno dei tre centri di distribuzione logistica. Nel quadro del piano industriale, pertanto, lo stabilimento di Stura, con la permanenza dell'attività di tessuti gommati tessili e metallici, manterrà la propria vocazione industriale, ed inoltre, con l'insediamento del Super Magazzino Amont e il trasferimento del magazzino di Vercelli, consentirà di occupare da 160 a 190 unità lavorative In data 1° dicembre 2008 è stato firmato il verbale di accordo tra la Michelin e le organizzazioni sindacali, in cui sono state previste le misure volte a fronteggiare i disagi causati allo stabilimento di Stura a seguito del citato piano di riorganizzazione. Tali misure si possono così riassumere: utilizzo, a partire dal mese di gennaio 2009, dello strumento della mobilità, sia per coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia durante la permanenza nelle liste di mobilità, sia per i lavoratori in esubero, riconoscendo loro delle integrazioni salariali; un piano sociale di incentivi finalizzato a sostenere la mobilità tra i siti. In particolare, per i lavoratori in esubero dello stabilimento di Stura che accetteranno di trasferirsi nello stabilimento di Cuneo, sono previsti incentivi per il pagamento dell'affitto, oltre al pagamento di una quota *una tantum* pari a 17.000 euro lordi; misure di accompagnamento finalizzate a sostenere i lavoratori che opereranno per soluzioni esterne, sia attraverso un programma di *outplacement*, sia attraverso misure di sostegno nei confronti di coloro che dovessero decidere di avviare una attività di impresa autonoma; la fase di transizione verrà gestita attraverso il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione a partire dal mese di luglio 2009. Il Ministero dello sviluppo economico seguirà, comunque, in modo attento l'evoluzione di questa vicenda, rendendosi disponibile fin da ora ad attivarsi su richiesta delle parti, al fine di affrontare le problematiche che dovessero emergere.

è vero che, secondo l'accordo, si tende a mantenere a Torino un'occupazione diretta, con almeno 350 posti di lavoro, in sinergia con Cuneo e che c'è anche un impegno a reindustrializzare l'area, in collaborazione con gli enti locali; ed è altrettanto vero che il potenziamento occupazionale produttivo del sito di Cuneo verso il mercato di alta gamma è uno degli obiettivi. Quindi, non soltanto la questione dei pneumatici fatti a Stura, ma il mercato di alta gamma a Cuneo

con la modalità di intergruppo (questi sono obiettivi necessari, ragionevoli, consueti) e con gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione straordinaria e mobilità esterna). Ed io apprezzo

riguarda il terreno del potenziamento e del coordinamento degli ammortizzatori sociali, è stato assunto l'impegno di fare tutto ciò che l'accordo prevede e forse anche qualcosa di più; e questo è senza dubbio apprezzabile. Quello che Quello che però voglio sottolineare è che, rispetto al 2 dicembre 2008, data dell'accordo, le cose sono ulteriormente peggiorate. Ora, non so se questo è dovuto ad un'aggressiva e crescente esportazione dei pneumatici prodotti in Estremo Oriente, ma sono comunque ulteriormente peggiorate. È previsto un incremento del ricorso alla cassa integrazione,

Questo porterà a riflessi occupazionali negativi specialmente ad Alessandria, e all'aumento della cassa integrazione ordinaria a Cuneo: Alessandria e Cuneo, quindi, sono ulteriormente colpite.

attivare quegli strumenti di politica industriale che possono consolidare l'occupazione e lo sviluppo produttivo di questa industria manifatturiera, che nell'indotto auto occupa, in Piemonte, 5.000 lavoratori.

oltre al mantenimento e allo sviluppo dello stabilimento di Stura, possa non vedere una polverizzazione della propria presenza in tutta la Regione Piemonte, trattandosi perlopiù di produzione di pneumatici del peso lordo, che riguardano i camion, i bus, eccetera. Quindi, vi è eccellenza, ma anche diffusione orizzontale di produzione.

lei, signor Sottosegretario, gestito dalla RAI in base ad una convenzione stipulata con lo Stato. La rete di diffusione Isoradio è di proprietà di una società controllata dalla RAI, la RAI Way, che sulla base della predetta convenzione Stato-RAI e compatibilmente con le risorse frequenziali a disposizione è tenuta a potenziare il servizio, sia in termini di copertura che di qualità di ricezione. In merito a quanto riferito dai senatori interroganti sulla qualità del servizio Isoradio, si fa presente che diverse sono state le difficoltà incontrate negli anni per porre a disposizione di tale servizio adeguate risorse frequenziali, per il mantenimento e il completamento della copertura nazionale. Isoradio presenta, infatti, vistosi scostamenti dalla unicità della frequenza, ad esempio nelle zone di Roma e Milano o in tratti toscani dell'autostrada Livorno-Genova, per preesistenti occupazioni private "sanate" dalla legge di disciplina n. 223 del 1990 (cosiddetta Tenuto conto che in molte zone del Paese la frequenza 103.3 è occupata da emittenti private, la RAI ha comunque provveduto ad ampliare la copertura territoriale di Isoradio acquisendo frequenze "limitrofe". L'estensione progressiva del servizio procede attraverso importanti interventi sulla rete di diffusione, svolti da RAI Way in collaborazione con i vari concessionari autostradali, l'ANAS e il Dipartimento della protezione civile. Si segnala a tale proposito la realizzazione della copertura continua di 260 chilometri dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, avvenuta nell'estate 2007 e ulteriormente migliorata nell'estate 2008. Ulteriori interventi tecnici hanno consentito la recente estensione della ricezione su ulteriori 110 chilometri di percorsi autostradali, principalmente sulla A1, A13 e A14, che permettono la ricezione del servizio Isoradio su oltre 3.000 chilometri di tratte autostradali. Attraverso il sistema RDS, ormai presente su tutte le autoradio, lo spostamento di frequenza avviene in modo automatico senza creare eccessivi disagi all'ascoltatore. Le informazioni trasmesse sulla viabilità provengono da Autostrade per l'Italia (in base ad una vecchia convenzione tra la RAI e la società Autostrade) e dalla Polizia stradale, attraverso due distinti sistemi informatici. Da quanto comunicato dalla RAI risulta che, a breve, i due sistemi saranno integrati e quindi sarà proprio la Polizia stradale, attraverso il CCISS-Viaggiare informati, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a gestire e a convalidare tutte le informazioni. Si ritiene, quindi, che il suggerimento proposto dalla senatrice Garavaglia di demandare al Dipartimento per la protezione civile la gestione dell'informazione sulla viabilità sia ormai superato dagli eventi, in quanto sarà la Polizia stradale a gestire la raccolta delle notizie sul traffico, mentre la RAI resterà il "vettore" principale per il loro inoltro su tutti i mezzi di comunicazione. In merito alla copertura della fascia oraria notturna in cui il servizio Isoradio è sospeso (dalle ore 00,40 alle ore 5,45), si segnala che le informazioni sulla viabilità vengono comunque trasmesse dalla RAI attraverso il canale Radio Per quanto riguarda, infine, il quesito relativo alle problematiche concernenti i contratti di lavoro degli operatori del Centro coordinamento sicurezza stradale e di Isoradio, si fa presente che il lavoro svolto da tali operatori della RAI è regolato dall'attuale contratto nazionale dei programmisti registi. A tale riguardo, la RAI ha precisato che taluni operatori hanno rivendicato in via giudiziale la novazione del contratto a giornalista professionista.

con piacere, come quello dell'unificazione informatica della presenza su molte nuove tratte. Rimangono però aperte alcune questioni. Intanto è importante che venga segnalata la possibilità, durante la notte, che è un momento abbastanza pericoloso sulle strade,

Signor Presidente, in relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue. L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), che fa capo attualmente alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia, dispone di un sito Internet che fornisce le informazioni relative alle concessioni di coltivazione ed ai permessi di ricerca di idrocarburi, al fine di rendere noti e accessibili i dati relativi all'attività di esplorazione petrolifera nel nostro Paese. Riguardo al recente "aggiornamento" del predetto sito, al quale fa riferimento il senatore interrogante, si precisa che il sito in questione non è stato oggetto di una nuova versione e che nello stesso non sono state inserite limitazioni di alcun tipo. Si precisa altresì che il sito, nella sua struttura consueta, viene continuamente aggiornato e migliorato. In relazione, poi, alle limitate opzioni del citato sito Internet, alle quali si fa riferimento nell'atto parlamentare in esame, si evidenzia che le carenze lamentate scaturiscono da una confusione tra i contenuti pubblicati, in particolare tra il collegamento «Titoli minerari vigenti» e il collegamento «Istanze per il conferimento di titoli Si tratta, infatti, di due basi di dati da sempre distinte, realizzate con finalità diverse e dotate di diverse funzionalità. Si fa inoltre presente tutte quelle funzionalità di cui si richiede il ripristino non sono mai state rimosse e sono tuttora presenti sul sito, dove è sempre possibile consultare l'elenco delle istanze per il conferimento dei titoli minerari per: eseguire ricerche mirate per Provincia, Regione e per richiedenti; visualizzare l'elenco delle coordinate geografiche dei vertici del poligono delimitante l'area richiesta; visualizzare la planimetria su tavola IGM alla scala 1 a 100.000; visualizzare in Google maps l'area interessata, sovrapposta ad immagini da satellite; monitorare l'*iter* relativo al conferimento, tramite la descrizione dei singoli passaggi effettuati e, in alcuni casi, visualizzando anche l'immagine del documento in formato pdf. Al riguardo, si precisa che le sopra citate caratteristiche sono proprie dell'elenco delle istanze e non sono mai state presenti nell'elenco dei titoli vigenti. Si precisa, altresì, che il sito Internet dell'UNMIG è visitato, quotidianamente, da numerosi utenti e che, grazie ai continui aggiornamenti, è ritenuto un fondamentale strumento di lavoro per gli operatori del settore e un utile strumento d'informazione per i cittadini. Si aggiunge, infine, che recentemente è stato sostituito il *server web* con una nuova macchina in grado di fornire il servizio con migliori prestazioni. L'ulteriore sviluppo del sito Internet consentirà, quindi, di rendere sempre più accessibili le informazioni dirette agli utenti.

diventa essenziale soprattutto per quelle realtà che vivono una condizione assai delicata, per l'impatto che le estrazioni petrolifere e minerarie determinano sul territorio. Pertanto, la mia preoccupazione, che mi permetto di affidare alla sua valutazione, è che gli strumenti di accesso siano il più possibile all'altezza di una larga condivisione. Da più parti, gli organi di informazione avevano sollecitato questa mia interrogazione, all'esigenza di ricevere una chiara informazione sia sui meccanismi amministrativi che regolano il settore, sia sullo stato dell'arte delle istanze. In una Regione come quella di mia elezione, la Basilicata, la presenza di istanze e di permessi di ricerca determina un coinvolgimento largo del territorio. È quindi utile avere contezza dall'Ufficio nazionale minerario dello stato delle cose. Mi permetto anche di rilevare che sarebbe il caso che l'Ufficio nazionale minerario, tramite i suoi strumenti di comunicazione, come il sito *web*, potesse dare anche informazioni puntuali su alcune questioni che sono altrettanto decisive, vale a dire la quantità delle estrazioni, che sono state oggetto spesso anche di controversia, le *royalties* maturate per i territori di estrazione e lo stato delle istanze, sia per la ricerca che per l'estrazione.